Presidente, desidero innanzitutto dichiarare che il Gruppo della Federazione della Libertà voterà contro il rendiconto e l'assestamento del bilancio al nostro esame. I provvedimenti che oggi esaminiamo non rappresentano un mero passaggio tecnico, o meglio si tratta di variazioni tecniche, magari sulle singole voci di bilancio, ma che

qui a valutare quali sono stati gli effetti delle politiche attive del Governo e quali alcuni degli effetti delle politiche in materia di riforme che sono state sbandierate sia, ovviamente, in sede nazionale,

Nonostante la lettura rosea dei dati che i colleghi relatori e gli esponenti della maggioranza hanno tentato di presentarci, noi crediamo che le politiche economiche di questo Governo e soprattutto il pesante lascito sui conti del precedente Governo Renzi non vadano nella direzione giusta. Riteniamo che il taglio della spesa abbia dato risultati deludenti e che le politiche di crescita siano state ancora troppo deboli e di corto respiro. Tutto questo, frutto soprattutto dell'azione di governo degli ultimi anni, ha creato ulteriore debito, portandolo a delle dimensioni abnormi e praticamente drammatiche. evidente che c'è la necessità di attivare politiche nuove, che diano un vero nuovo slancio al Paese. al Paese. I temi sono tanti e li abbiamo discussi a fondo in occasione dell'esame della legge di bilancio e delle manovre correttive e proprio per questi motivi riteniamo che ci debba essere uno slancio maggiore in termini di proposta

Questo rendiconto e questo assestamento dimostrano la debolezza delle politiche che sono state attivate fino ad oggi e pertanto il Gruppo della Federazione della libertà esprimerà voto contrario.

Governo e dei Governi che si sono susseguiti in modo più o meno legittimo dal 2011 ad oggi. Dico più o meno legittimo perché sono stati frutto di scelte non compiute dai cittadini con un voto democratico, ma esclusivamente con l'appoggio di Gruppi parlamentari che si sono uniti in queste Aule, non necessariamente su un progetto politico o su una linea di governo voluta e votata dai cittadini, ma esclusivamente per portare avanti questa legislatura e quella precedente. e quella precedente. I Governi che si sono succeduti - da Monti a Letta, a Renzi ed oggi a Gentiloni Silveri - hanno attuato sostanzialmente due tipi di scelte e di politiche economiche: all'inizio, con il Governo Monti, la strategia dell'aggressione nei confronti dei risparmi dei cittadini italiani, con azioni basate sull'aumento della pressione fiscale anche in modo sconsiderato, deprimendo l'economia. Questa è stata la prima cura che, di fatto, ha danneggiato in modo irreversibile la qualità e la forza trainante dell'economia del nostro Paese, in particolare dei territori del Nord, distruggendo il sistema manifatturiero che si creato con grande fatica. Poi c'è stata la politica renziana, quella dei *bonus*, quella di una spesa che non ha prodotto sviluppo economico, ma che è andata esclusivamente alla ricerca di un continuo consenso elettorale che poi è svanito nella notte del 4 dicembre con una bocciatura perentoria e senza appello da parte dei cittadini italiani.

che portano a risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che, in modo anche abbastanza ridicolo, l'attuale Governo vuole presentare come miglioramenti dell'economia in una situazione sotto controllo che di fatto non esiste. nel momento in cui il Governo, attraverso la relazione che è stata svolta in questa sede, ma anche attraverso la propaganda che viene proposta sugli organi di informazione, afferma che abbiamo agganciato la ripresa, che il PIL cresce e che quindi, siamo fuori dalla crisi, dà notizie assolutamente prive di fondamento perché a fronte di un aumento del prodotto interno lordo italiano che è

apparente e dovuta ad una situazione momentanea - e non quindi strutturale - positiva a livello internazionale. I dati, quindi, mostrano una assoluta bocciatura,

ma anche perché nei dati di fatto, per la realtà che noi viviamo nel Paese tutti i giorni, non avvertiamo la ripresa di cui si narra e di cui si vogliono illudere i cittadini italiani. Noi ravvisiamo ancora, sul nostro territorio, per chi vive la realtà del nostro territorio, situazioni di crisi delle famiglie, delle imprese, delle attività commerciali e artigianali che aprono e chiudono continuamente nel giro di pochi mesi proprio perché ormai intraprendere attività nel nostro Paese è praticamente impossibile. Siamo in questa situazione e siamo in una situazione ancora più assurda e aberrante perché, a fronte di una politica di questo tipo, noi assistiamo ad una continua fuga da parte di cittadini italiani all'estero. Questo è un dato che non viene rilevato da queste analisi macroeconomiche, ma che per noi ha una valenza fondamentale. Noi abbiamo assistito, nel 2016 e negli anni precedenti, ad un continuo arrivo di extracomunitari; in particolare l'anno scorso sono stati oltre 170.000. Si tratta di non di rifugio, non di un luogo dove non esiste la guerra, ma semplicemente di un luogo dove costruire un futuro economico per se stessi, a fronte di 110.000 italiani che sono emigrati. Questi dati dovrebbero preoccupare il Parlamento e il Governo perché rappresentano un modello assolutamente

nel suo testo originario, stanzia, in aggiunta a quelli già previsti, 600 milioni per le politiche a favore degli stranieri, dei richiedenti asilo e dei profughi e altri 134 milioni per politiche connesse al permesso di soggiorno e alla qualifica dei rifugiati.

di persone con disabilità, non autosufficienti e invalidi civili e di 50 milioni per le politiche della famiglia. Questo è l'emblema della politica economica del Governo: una spesa incontrollata per l'ospitalità e per favorire l'ingresso di extracomunitari e di manodopera a basso costo, dall'altra un taglio della spesa destinata alle fasce deboli della nostra popolazione.

manodopera a basso costo e alterare l'identità dei nostri popoli e delle nostre comunità, perché è evidente che è più facile dominare popoli senza identità, piuttosto che popoli che abbiano un identità forte e gli strumenti per difendersi dai poteri forti, dalla dall'arroganza della politica. È un modello sociale al quale non ci rassegneremo. È un modello di sviluppo del futuro del nostro Paese e dei nostri territori al quale non ci vogliamo adeguare, che riteniamo sbagliato e che non consideriamo inevitabile. Anzi, Anzi, riteniamo che sia un modello voluto, pianificato, studiato e finanziato da questo Governo e da altri Esecutivi di questo genere, che rappresentano un sistema di potere che non identifica nei cittadini individui che hanno diritti, ma esclusivamente consumatori, persone che devono produrre e pagare.

L'aspetto peggiore di tutta questa vicenda è che ciò sta accadendo ormai nella totale indifferenza del Governo e nella totale rassegnazione dell'opinione pubblica italiana. Noi diciamo no a questi provvedimenti economici per tutti i motivi che ho esposto e per le politiche alle quali sottende la spesa di questo Governo. Diciamo no perché rappresentiamo una forza politica che non si rassegna

manifesta forme di incompletezza e approssimazione e la presenza di norme *spot*, scollegate tra loro e totalmente inutili a fare immaginare una qualsivoglia forma di ripresa e non fa altro che aggravare un quadro economico già di per sé disastroso. Faccio una previsione: quando questo Governo il prossimo anno finirà il suo mandato, il debito pubblico raggiungerà i 2.500 miliardi. Valutando l'aspetto delle spese in conto corrente e in conto capitale, ci si rende immediatamente conto di come queste ultime siano sempre poche e ridotte, quando in realtà sono proprio quelle che nel lungo periodo danno un ritorno positivo in termini di lavoro, occupazione e, più in generale, in favore della crescita economica.

politiche di svecchiamento nella pubblica istruzione: nelle nostre scuole abbiamo bisogno di giovani più preparati che sostituiscano il personale ultrasessantenne - chi vi parla ha quella età che ormai non ha più motivazioni, non fa più aggiornamento e non è più in grado di formare il futuro quadro lavorativo del Paese.

perché se questi entrano nelle forze sanitarie produttive ci può essere ripresa. Sono queste le riforme strutturali; è questo l'uovo di Colombo e il coraggio che negli anni Ottanta ha avuto Bettino Craxi quando siamo diventati la quinta potenza economica mondiale. Di contro, ad aggravare ulteriormente questo contesto già compromesso, la spesa corrente continua a risentire di una *spending review* poco efficace, perché poco seria, in quanto basata esclusivamente su tagli lineari. sono utili solamente a buttare fumo negli occhi ai cittadini al fine di cavalcare l'onda sempre più lunga del populismo. Si tratta di una strategia utile forse in termini elettorali, ma che comunque non potrà durare ancora a lungo, sia perché inconcludente, sia perché i benefici derivanti dai tagli ai costi della democrazia sono irrisori almeno quanto i costi stessi. Bisogna, innanzitutto, puntare a incrementare le entrate, perché solo in questo modo si potrà recuperare il terreno perduto in questi anni per cause dovute sia al contesto economico internazionale che a fattori esclusivamente interni. È necessario comprimere il *gap* tra le varie fasce della popolazione e ancor più urgente è puntare a smussare quella differenza ancora troppo netta tra il Nord e il Sud del Paese, un antico e dannoso retaggio che è giunta l'ora di superare. Colleghi, questo non lo si fa con gli *spot* preelettorali o con tagli che non incidono per nulla sul bilancio dello Stato. Il medico non può garantire con le sue cure la vita eterna. Anche in questo caso c'è necessità di essere pragmatici di non dire che va tutto bene quando non si fanno le riforme strutturali e quando sugli investimenti non si puntano quantità di denaro tali da permettere lo sviluppo stesso in ricerca e innovazione. Siamo stati una Patria che ha insegnato al mondo le nostre capacità nel terziario avanzato e dobbiamo cercare non di tagliare, ma di investire quanto più possibile Certo, controllo e contenimento della spesa pubblica devono essere posti tra le priorità, ma è necessario soprattutto puntare a rilanciare i consumi e gli investimenti, sostenendo la semplificazione, riducendo la pressione fiscale, abbandonando forme di assistenzialismo, assistenzialismo, incentivando la giustizia sociale e favorendo un processo di riforme strutturali serie. Colleghi, la malagiustizia e la medicina difensiva ci costano dai 20 ai 40 miliardi,

Insomma, invece di galleggiare servendosi di annunci e proclami, urge rimettere effettivamente in moto la nostra economia e occorre che questa giunga quanto prima a pieno regime. Per fare ciò serve incidere anche con investimenti che potremmo definire di carattere culturale, puntando a far emergere il cosiddetto sommerso e incentivando la cultura della legalità tanto nel mondo del lavoro che in quello imprenditoriale. Per fare questo, non basta tagliare. Tagliare gli sprechi è doveroso, moralmente obbligatorio, ma quello che conta finanziariamente è investire e investire bene, puntando al rilancio di quelle aree nelle quali il tasso di povertà e di disoccupazione ha una percentuale maggiore e indirizzandosi effettivamente sulle nostre eccellenze, anche intellettuali, decantate ovunque nel mondo, come dicevo prima. Il quadro economico, che rispetto a qualche anno fa ci appare leggermente migliore, non deve ingannarci, così come la lettura e la conseguente analisi dei dati ISTAT non devono essere un mezzo per fare propaganda. I dati vanno, infatti, letti tutti nel loro complesso, interconnettendoli tra loro. Tasso di occupazione e volume dei consumi, ad esempio, sono strettamente collegati e non basta che solo uno dei due abbia un indice positivo per illudersi che vada tutto bene. È per questo che pongo nuovamente l'accento sull'esigenza di superare una facile leggerezza quando si stende e si esamina questo tipo di provvedimenti ed invito il Governo e la maggioranza ad abbandonare la ricerca del consenso al di fuori delle Aule parlamentari e a puntare a una crescita effettiva e sostanziale,

questo nell'economia e nello sviluppo del Paese non abbiamo bisogno. Questo coraggio, a noi del Gruppo Ala-Scelta Civica, è sembrato totalmente assente nell'intero ciclo che riguarda i provvedimenti economici sottoposti al vaglio del Parlamento. Dichiaro,

Signora Presidente, onorevoli senatori, da sempre la valutazione del rendiconto generale dello Stato nelle Aule parlamentari risponde alla funzione giuridico-costituzionale di controllo del Parlamento sull'operato dell'Esecutivo, per verificare se il Governo abbia dato seguito in modo corretto alla gestione finanziaria nei termini preventivamente stabiliti mediante l'approvazione della legge di bilancio annuale. La struttura dell'intero atto si presenta pertanto come molto complessa e tecnica, comprendendo infatti il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. In particolare, il conto generale del patrimonio risulta essere il documento contabile in grado di presentare la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio per effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e passivi

con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era invece assestato ad un valore negativo di 41,5 miliardi. Il risparmio pubblico nel 2016 evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente, assestandosi a più 32,8 miliardi, a causa sia dell'aumento delle entrate correnti (più 16,7 miliardi), sia della diminuzione della spesa corrente (meno 20,2 miliardi). Nel documento economico-contabile si conferma poi un dato già noto: nel 2016 il PIL ai prezzi di mercato registra una crescita nominale dello 1,6 per cento rispetto all'anno precedente e una variazione in volume anch'essa di segno positivo pari allo 0,9 per cento, confermando un dato in crescita quasi identico a quello registratosi nel 2015 (0,8 Tuttavia, qui mi preme fare una valutazione politica, perché non possiamo non registrare che a dieci anni dalla crisi, il PIL italiano è stimato ancora a livelli inferiori di quello del 2007 di circa otto punti, con una perdita cumulata di circa 800 miliardi di euro. I problemi investono sia il lato della domanda (consumi inferiori del 5 per cento, investimenti di quasi il 30 per cento), sia il lato dell'offerta con una perdita ulteriore di produttività del lavoro. Questi numeri sono il segno di politiche economiche sbagliate ed inefficaci, perché se si continua a seguire una politica dell'offerta basata sulla contestuale riduzione della spesa e delle imposte

In connessione funzionale con lo strumento del rendiconto di bilancio, bisogna procedere all'esame del disegno di legge di assestamento 2017, che, nel configurarsi come il primo a essere predisposto conformemente alle più recenti modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si conferma un atto non solo necessario, ma fortemente opportuno per mettere a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni. È vero che il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a 17,4 miliardi. Tuttavia, occorre sottolineare che il valore è comunque coerente con il limite massimo stabilito dall'allegato 1 dalla legge di bilancio 2017 come successivamente modificata. Si accoglie favorevolmente il risultato dell'aumento delle entrate per 2,8 miliardi e della riduzione della spesa per interessi per 1,9 miliardi. Altrettanto favorevolmente si registra il dato per cui le previsioni circa il risparmio pubblico migliorano rispetto a quelle iniziali per un valore di 2,9 miliardi. Bene anche il dato sulle entrate finali che aumentano di 5,3 miliardi rispetto alle previsioni, frutto di un incremento delle entrate tributarie per 1,8 miliardi e di quelle extra-tributarie per 3,5 miliardi. È importante evidenziare poi come le proposte di assestamento formulate con il presente disegno di legge migliorano i saldi di finanza pubblica, sia aumentando le entrate di 2,8 miliardi, sia con una riduzione delle spese finali per 1,6 miliardi imputabile alla rilevante riduzione della spesa per interessi, sia riducendo il rimborso delle passività finanziarie. Il quadro economico si assesta con queste condizioni perché, purtroppo, si registra un peggioramento dell'avanzo primario e le previsioni assestate delle spese finali fanno registrare un incremento di 22,7 miliardi, tanto al livello di spese correnti, quanto al livello di spesa in conto capitale. Il Gruppo Articolo 1-Movimento Democratico Progressista voterà dunque a favore di questi provvedimenti. Signora Presidente, l'esame del rendiconto generale dello Stato in sede parlamentare riflette la funzione giuridico-costituzionale di controllo del Parlamento sull'Esecutivo, rappresentando lo strumento attraverso il quale si verifica che il Governo abbia dato effettivo seguito alla gestione finanziaria nei termini preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento, mediante l'approvazione della legge di bilancio annuale. Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, si registra un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive come risultanti dalla legge di assestamento 2016, sia rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015. In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2016 presenta un valore negativo pari a 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era invece assestato ad un valore negativo di 41,5 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è risultato migliore di 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di 38,9 miliardi di euro. Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 42,8 miliardi, il rendiconto 2016 segnala un lieve aumento rispetto all'anno precedente di 1,5 miliardi, che fa ben sperare per l'aumento degli investimenti in futuro, legato in particolare alla ripresa del ciclo economico.

Le proposte di assestamento formulate con l'altro disegno di legge in esame oggi in quest'Aula per l'esercizio finanziario 2017 migliorano i saldi di finanza pubblica sia aumentando le entrate (+2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (1,6 miliardi) e il rimborso delle passività finanziarie (5 miliardi). Con riferimento alle spese finali, la riduzione di 1,65 miliardi è imputabile alla consistente riduzione della spesa per interessi per 1,95 miliardi di euro, che attenua l'aumento di 253 milioni della spesa corrente al netto degli interessi e di 45 milioni della spesa in conto capitale. Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi ad eccezione del risparmio pubblico. L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 20 miliardi (dai circa 102,6 miliardi delle previsioni iniziali a 122,6 miliardi),

23,4 miliardi, giunge a un importo ugualmente negativo di poco meno di 45,7 miliardi, con un peggioramento percentuale di poco inferiore al 96 Il solo risparmio pubblico migliora di 3,3 miliardi, passando da circa 61,2 miliardi a circa 57,9 miliardi. Degna di nota invece la differenza di quasi 2,7 miliardi di euro tra la consistenza delle spese finali in termini di competenza e di quelle in termini di cassa, spiegata dallo smaltimento dei residui passivi. La composizione delle variazioni formulate dall'assestamento, articolate per missioni, mette in evidenza tra le variazioni più significative: la minore necessità di rimborso di prestiti internazionali, con una riduzione della missione Debito pubblico pari a 6,15 miliardi in termini di competenza e 6,4 miliardi in termini di cassa;

la riduzione di spesa delle Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali pari a circa 1 miliardo in termini di competenza (841 milioni in termini di cassa), dovuta principalmente alle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a Statuto speciale,

e ai connessi trattamenti di fine rapporto; l'incremento di 990 milioni (solo in termini di cassa) della missione Soccorso civile in seguito alle assegnazioni in favore degli uffici speciali a L'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione; infine un aumento di oltre 550 milioni (competenza e cassa) relativi a Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, dovuto al maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori. Dall'esame pur breve dei principali macrodati emerge un elemento significativo: il nostro Paese è in ripresa costante. L'azione del Governo e di questo Parlamento, seppur difficoltosa per la congiuntura economica a livello internazionale, in questi cinque anni ha dimostrato la capacità del Paese di rialzare la testa e di guardare con ottimismo al futuro. Chiaramente non siamo soddisfatti, in quanto questi dati in ripresa devono essere unicamente un primo stimolo per migliorare ulteriormente il quadro generale del sistema Paese. azione macroeconomica della maggioranza non potrà che sostenere ulteriormente la crescita, incentivando le spese in conto capitale, foriere di ricadute positive in termini occupazionali e di gettito erariale. Le spese per il sostegno del lavoro non potranno certamente diminuire, ma al tempo stesso bisognerà cercare le modalità per aumentare ulteriormente gli sgravi fiscali agli imprenditori, al fine di sostenere ulteriori assunzioni. Soprattutto la programmazione dell'innovazione infrastrutturale dovrà assumere i caratteri della sistematicità. fermo agli anni Sessanta per tanti aspetti, non può più prescindere da una corretta gestione del proprio territorio e, anche alla luce dei cambiamenti climatici, dovrà dotarsi di un piano di gestione delle acque, di contrasto al dissesto idrogeologico in generale e di una mappatura sismica seria dell'intero Stivale. Se non iniziamo a stanziare somme sistematiche su questi aspetti, ritroveremo nel tempo a rincorrere costantemente le emergenze e a rattoppare ciò che non è più rattoppabile, ma che va drasticamente mutato.

in particolare, prevede un peggioramento del saldo netto da finanziare di 21,9 miliardi per atti amministrativi. Tradotto, si tratta dell'impatto di 20 miliardi di euro su tale saldo 237 del 2016, cosiddetto salva banche, che ha comportato un incremento delle acquisizioni di attività finanziarie per tale somma. L'assestamento è stato poi aiutato, per così dire, dalla riduzione della spesa per interessi per circa 2 miliardi e dall'aumento delle entrate per circa 3 miliardi dovuto alla ripresina in corso. Le spese sono state ridotte di circa un miliardo. Alla fine, il saldo netto da finanziare peggiora in termini di competenza di 17,4 miliardi rispetto al dato indicato nella legge di bilancio per il 2017. Insomma, quando si tratta di finanziare gli istituti di credito non si bada a spese, non ci si preoccupa dei saldi di finanza pubblica. Tutt'altra musica, invece, per la sanità, la scuola, le pensioni, il contrasto dei cambiamenti climatici e l'intervento per la cura del territorio. Con gli ultimi emendamenti presentati ieri dal Governo si finanziano ulteriormente, di 100 milioni, le spese generali del Ministero della difesa, mentre per dare altri 18 milioni ai nostri servizi di informazione non si trova niente di meglio che toglierli alla cooperazione migratoria. Meno male che lo *slogan* di quest'estate era: «Aiutiamoli a casa loro». Il voto su questo provvedimento e sul rendiconto 2016 esprime a nostro avviso un giudizio più generale sulle politiche di finanza pubblica di questo Governo e del precedente Il Governo si gloria della maggior crescita attuale. Vorrei riportare al riguardo alcune osservazioni dell'ex responsabile dell'ufficio studi di Bankitalia, Pierluigi Ciocca: «Questi sono i dati di una ripresa ciclica non consolidata nelle componenti della domanda, e mediocre, sia in assoluto sia nel confronto internazionale. Soprattutto, mediocre rispetto a un crollo che dai picchi ciclici trimestrali di dieci anni fa

Si ha crescita quando la progressione del prodotto, oltre a essere tendenziale (non ciclica), più che da un maggiore impiego del lavoro e delle altre risorse già disponibili ma sottoutilizzate, scaturisce principalmente da una intensificata accumulazione

per poi precipitare al 6,4 per cento nel 2019, lasciando intendere che l'eventuale ripresa del PIL non avrà ricadute in alcun modo positive sul finanziamento pubblico della sanità La Corte dei conti quantifica che nel periodo 2015-2018 l'attuazione degli obiettivi di finanza pubblica ha determinato una riduzione cumulativa del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 10,51 miliardi di euro, rispetto ai livelli programmati.

Altro elemento di riflessione riguarda le spese militari e in particolare il programma di acquisizione degli F-35. Un programma originariamente previsto in più di 18 miliardi che, sempre secondo la Corte dei conti, ha visto raddoppiati i costi unitari ha avuto un impatto occupazionale molto ridotto anche rispetto alle stesse previsioni iniziali. È stata bocciata anche la modesta proposta dell'onorevole Damiano, presidente della Commissione lavoro della Camera, di bloccare l'aumento dell'età pensionabile, in particolare per le donne. La più alta in Europa. Niente da fare, i tagli al *welfare* devono proseguire. Dunque, due pesi e due misure. Il Governo, con la presentazione della Nota di aggiornamento del DEF (tra qualche giorno), si appresta a chiedere al Parlamento la deroga dal percorso di avvicinamento verso «l'obiettivo di medio periodo» (il pareggio di bilancio). Non è la prima volta. Anzi, se non vado errata, si tratta della quinta volta che ciò accade. La cosa ha un che di surreale, avendo il Parlamento tutto, nella scorsa legislatura, approvato una modifica dell'articolo 81 della nostra Costituzione che costituzionalizzava, per l'appunto, il pareggio di bilancio. Come Sinistra italiana non solo abbiamo presentato una proposta di modifica di tale norma, ma nel corso dell'*iter* della riforma costituzionale renziana, abbiamo presentato un emendamento in tal senso che è stato ovviamente respinto dalla maggioranza; maggioranza che oggi chiede un voto trasversale per derogare dalla norma che essa stessa ha fortemente voluto e voluto mantenere in Costituzione. Non saranno alcune parziali proposte correttive alla prossima legge di bilancio che determineranno una reale discontinuità con le politiche di austerità espansiva perseguite da questo Governo. Serve una reale correzione di rotta rispetto Renzi ha proposto di portare il *deficit* per cinque anni vicino al 3 per cento, ma poi ha subito precisato che si tratta di un programma per la prossima legislatura

Non condividiamo poi l'utilizzo che continua ad essere proposto, anche in vista della prossima legge di bilancio, di questa maggiore flessibilità di bilancio: la moltiplicazione di inutili *bonus* che, come si è visto dall'esperienza di questi quattro anni, non hanno certamente avuto un positivo effetto moltiplicatore. Serve una politica di investimenti pubblici dedicata alla conversione ecologica del nostro sistema produttivo, a rimediare al dissesto idrogeologico del nostro Paese, alla messa in sicurezza antisismica e a un vero e proprio piano di adattamento ai cambiamenti climatici, dando così lavoro qualificato a centinaia di migliaia di giovani. Francia e Germania mascherano i loro interessi nazionali sotto presunti ideali europeisti. L'Italia deve saper difendere i propri interessi nazionali e pesare in Europa. Il nostro Paese può gettare tutto il suo peso nella riforma del *fiscal compact*, che dovrebbe essere inserito entro quest'anno nei Trattati europei. Bisogna avere il coraggio di farlo, pena la riduzione del nostro Paese

per molti aspetti ho avuto la sensazione di riascoltare sempre la solita propaganda, come quando si scrivono i *tweet* e si fa il solito gioco con i numeri,

Perché dico questo? Perché, ogni volta, c'è un autoincensarsi, soprattutto da parte dell'elegante ex *Premier,* ora segretario del Partito Democratico,

quindi mese con mese. Allora, se a giugno abbiamo avuto un +1,1, che è un dato significativo, un incremento deciso che che ha portato un buon contributo alla produzione industriale (ma bisogna considerare anche la componente energetica perché, volenti o nolenti, è così, signori, e basta andare a leggere anche il rapporto Terna per sapere il perché), arriviamo a luglio e la crescita congiunturale, ossia mese su mese, è dello 0,1

il dato 2010, che è l'anno di riferimento, siamo a 96,9. Quindi, siamo ancora distanti però stiamo cercando di avvicinarci al 100 del 2010. Ma se guardiamo un po' tutta la progressione, vediamo che a dicembre 2016 - e di questo devo rendere merito, purtroppo, a Renzi - eravamo già a 96,2, e a gennaio c'è stata una contrazione decisiva e poi c'è stata una contrazione in aprile che ci aveva portato a 94.

l'aumento del debito pubblico: il debito pubblico galoppa e il PIL affanna rispetto al debito pubblico. Questo è sbagliato, è una distorsione che bisogna evidenziare, perché altrimenti non si va avanti.

perché, in realtà, c'è il *quantitative easing* che ci ha fatto risparmiare 10 miliardi di euro di interessi passivi e non è un'azione del Governo e c'è un taglio feroce a carico delle amministrazioni locali, pagano il debito, quando invece quello delle amministrazioni centrali non fa altro che aumentare. E qui veniamo al sentiero stretto di cui ha parlato il vice ministro Morando.

arriva dal Governo Renzi, che, dopo le clausole di salvaguardia del Governo Letta di 3, 7 e 10 miliardi, arriva quasi a 30 miliardi di clausole di salvaguardia: sono quegli aumenti dell'IVA e delle accise che non ci permettono di agganciare la vera crescita, quella europea. Se ci andrà bene, all'Italia toccherà una crescita dell'1,5 per cento contro una media del resto d'Europa del 2,2. Noi siamo sempre dietro,

inutile che twittate sul rapporto della BCE: leggetelo bene. È una spesa fatta a *deficit*, che ancora dobbiamo saldare e che ancora oggi non ci consente di dare man forte neanche a quella produzione industriale fatta con gli sgravi, perché anche quella è una norma *spot*, è una droga, come ha detto il vice ministro ministro Morando. Non ci permette di andare oltre e di quei 10 miliardi spesi solo 3,5 miliardi sono stati spesi al consumo e questo è un dato agghiacciante, preoccupante: non c'è niente di cui essere contenti rispetto Adesso siamo qui ad incartarci per cercare un miliardo o 1,5 miliardi per prorogare gli iperammortamenti, norma *spot*,

per il fatto che sono stati spesi male i soldi, per il fatto che magari nell'evasione fiscale, nella semplificazione, c'è stata una serie di avvicendamenti di proroghe su scadenze già trascorse, dove è stata magnificata la vostra incompetenza - e le aziende, le imprese ed i professionisti che in questi giorni hanno a che fare con questi rinvii e con la comunicazione dei dati IVA sanno benissimo di cosa sto parlando e mi auguro che se ne ricordino quando sarà il momento - noi voteremo no a questo rendiconto, per una questione di maturità e di responsabilità e perché i numeri noi li leggiamo tutti e per bene.

sulle ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà contro l'assestamento di bilancio che oggi ci viene presentato. Non vi è dubbio che

portati dalla legge di assestamento, si capisce che la situazione della finanza pubblica italiana non è sotto controllo. Si è già detto che

in termini di competenza per 17,4 miliardi e ciò è molto grave, ma è ancora più grave perché peggiora di più in termini di cassa il peggioramento della cassa rispetto alla competenza continua ad indicare una spesa corrente che aumenta ed è fuori controllo. Questo è il dato di fondo che emerge da questo bilancio

peggiora il ricorso al mercato, che è naturalmente la differenza tra le entrate finali ed il totale delle spese e quindi significa che dovremo ricorrere all'emissione di titoli e dunque al debito. Soprattutto, peggiora l'avanzo primario: tutti tutti ricordano che tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del 2000, una bandiera del centrosinistra era quella di aver migliorato l'avanzo primario. Non è qui il caso di vedere perché allora migliorò, ma ma intanto questo era ritenuto uno dei segnali di buona finanza pubblica. Bene: l'avanzo primario peggiora, addirittura

di migliorare il rapporto debito-PIL che è quanto oggi ci chiede l'Europa ma soprattutto è la vera zavorra che frena che frena le possibilità di sviluppo in Italia. L'avanzo primario diminuisce. Vi è un altro dato che sembra migliore, cioè quello del risparmio pubblico, è la differenza tra le entrate correnti e le spese correnti al lordo degli interessi pagati. Si capisce che il risparmio pubblico migliora perché il tasso degli il tasso degli interessi sul debito pubblico è in assoluto, in maniera straordinaria, più basso rispetto a tutto il periodo precedente, almeno a mia memoria. questa favorevole congiuntura seppure fa migliorare il risparmio pubblico, come ho detto prima, non è però capace di migliorare l'avanzo primario ed ecco perché il quadro è francamente e certamente negativo. Naturalmente, che incrementino le spese correnti è un dato importante. aumentano nell'ordine di quasi 3 miliardi di euro: questo significa che abbiamo ancora una situazione della spesa corrente che non è sotto controllo. E, quasi beffardamente, signora Presidente e colleghi, sembra che aumentino le spese in conto capitale

relative agli investimenti. No: viene considerata spesa in conto capitale anche l'acquisizione di attività finanziarie. Ed ecco l'aumento di 20 miliardi perché, come sapete, sono stati necessari 20

Ed allora è sufficiente, come diceva stamattina il vice ministro Morando, quel sentiero stretto per rimettere in piedi l'Italia? No. Io credo che non sia possibile. C'è bisogno, invece, più che di un sentiero stretto di una veduta larga, di un vero cambiamento di rotta, di un Governo che abbia il coraggio di fare alcune cose importanti che limitino grandemente la spesa corrente e diano agli investimenti pubblici, che sono compito del Governo, un significativo aumento. È vero, sono d'accordo con il vice ministro Morando sul fatto che l'insieme delle misure per le industrie - ammortamenti, crediti d'imposta ed altro - sono state, in questo momento, degli elementi positivi, che hanno in un certo modo contribuito alla ripresa che in questi mesi si sta verificando, ma, attenzione, ci sono molti indicatori che dicono che l'attuale ripresa non ha carattere strutturale e comunque la nostra ripresa è largamente inferiore a quella dei nostri *competitor* europei. Allora perché sono necessari una un cambiamento di rotta? Faccio solo un esempio, relativo agli investimenti pubblici. C'è un grafico che mette i brividi in chiunque lo legga: nel 2016 le somme appostate per gli investimenti pubblici sono state di gran lunga maggiori che negli anni precedenti, ma le somme spese sono state di gran lunga minori, addirittura addirittura in valore assoluto, rispetto a quelle precedenti. Ed ecco la veduta larga: non è che forse quel complicatissimo meccanismo del nuovo codice degli appalti, che si sussegue a quello precedente e che non si sa come vi si sovrappone, è davvero uno degli elementi che frena il tradursi dell'appostamento di bilancio in investimento concreto e quindi in occupazione, lavoro e ricchezza? Non è che quel profluvio di autorità, semiautorità e ultrautorità, che riteniamo debbano dare una patente di legittimità a tutto, in realtà

complesso di economie esterne che favoriscano gli investimenti pubblici, quelli privati e contribuiscano ad attrarre quelli esteri. Solo questo può contribuire seriamente alla ripresa dello sviluppo in Italia in maniera strutturale. Con quel sentiero stretto e queste manovre di assestamento, che denotano ancora un uso largheggiante di spesa corrente rispetto alle necessità di una finanza pubblica sana e che promuova invece esclusivamente lo sviluppo, non ci siamo non ci siamo proprio. Ed è per questo che il Gruppo di Forza Italia voterà contro la proposta di assestamento. *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento di assestamento del bilancio pubblico per l'anno 2017 rappresenta un passaggio importante del ciclo di bilancio. In questa circostanza esso giunge a proposito per confermare a tutti noi e ai nostri concittadini, che l'Italia ha i conti pubblici in controllo e un'economia che finalmente mostra segni significativi di ripresa. Gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT confermano che il Paese si trova oggi nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente. Sul fronte della finanza pubblica, l'assestamento 2017 ci conferma che il *deficit* pubblico è sotto controllo e l'avanzo primario, pur in diminuzione, è tutt'ora fra i diminuzione, è tutt'ora fra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione europea. Questo è bene ricordarlo. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, risulta pari a circa 56 miliardi di euro con un peggioramento di circa 17 miliardi rispetto al dato indicato nel disegno di legge di bilancio 2017 (38,6 miliardi). Dal lato delle entrate le proposte di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa un miliardo di euro, ma vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare. Per quanto riguarda le entrate finali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto a quelle iniziali, come risultato di un incremento delle entrate tributarie e di quelle extratributarie. Rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2017, si evidenzia un netto miglioramento del risparmio pubblico. Le proposte di assestamento formulate con il disegno di legge in esame e gli emendamenti approvati migliorano i saldi di finanza pubblica sia aumentando le entrate sia riducendo le spese finali e il rimborso delle passività finanziarie. Alla luce dei dati sintetici ricordati, si conferma la sostanziale tenuta dei nostri conti pubblici e soprattutto la ritrovata credibilità internazionale del Paese, che si riflette nella positiva caduta dei tassi d'interesse sui titoli del nostro debito pubblico. Lo *spread* non rappresenta più un elemento di tensione, di instabilità e di caduta della fiducia nei confronti del nostro Paese. Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali internazionali con una situazione di finanza pubblica credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari internazionali. Ma il dato maggiormente positivo di questi mesi è che l'economia nazionale si sta avviando verso una decisa ripresa economica e occupazionale. Nelle scorse settimane, l'ISTAT ha diffuso una serie di dati confortanti: il prodotto interno lordo ha registrato nel secondo trimestre dell'anno in corso una crescita pari allo 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,5 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2014.

percentuali alla crescita del PIL. Anche la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del PIL (+0,1 punti percentuali). Alcuni affermano che è poco - lo abbiamo sentito anche in questa discussione - ma certo non si può negare che sia il quarto trimestre consecutivo in cui si registra una variazione tendenziale positiva dopo la caduta registrata tra il primo e il secondo trimestre del 2016. È un *trend* di crescita ormai consolidato

L'incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno - è importante - e l'occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria. La crescita dell'occupazione riguarda entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è più intensa per le donne e nel Nord. A conferma del buon andamento del mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,6 punti in confronto a un anno prima, con maggiore intensità per quello giovanile. L'inflazione si attesta su livelli lievemente positivi. Il ritmo di crescita annuo dell'indice per l'intera collettività (NIC) risulta dello 0,3 per cento su base mensile e dell'1,2 per cento rispetto ad agosto 2016.

Secondo il Fondo monetario internazionale, i dati relativi al secondo trimestre mostrano che nell'area euro l'Italia è cresciuta più del previsto. Un Paese in queste condizioni economiche, sociali e di finanza pubblica, pur ancora difficili, può guardare al futuro con maggiore fiducia rispetto Non esistono bacchette magiche per la crescita economica, ma dobbiamo ricordare le difficoltà affrontate nei primi provvedimenti esaminati all'inizio di questa legislatura. Eravamo in una situazione di stagnazione economica completa con tutti segni negativi con dati occupazionali di emergenza. Il mondo delle imprese era in forte difficoltà. La stretta creditizia e l'incertezza dei mercati finanziari dominavano la scena e condizionavano le scelte di politica economica. Il nostro Paese era osservato speciale in Europa e dovevamo affrontare manovre su manovre per portare i conti sotto controllo. oggi con orgoglio possiamo dire che il duro lavoro fatto in questi anni dai nostri Governi e dalla maggioranza che li ha sostenuti è stato positivo. Le scelte adottate sono state la giusta ricetta per far ripartire il Paese. Il Governo Renzi ha varato importanti misure che sono state alla base del *trend* di crescita che oggi registriamo, come ad esempio il tanto discusso aumento mensile di 80 euro per 11 milioni di lavoratori, che proprio ieri le istituzioni europee hanno giudicato *a posteriori* come un provvedimento fondamentale per il rilancio dei consumi e del PIL del nostro Paese. Non posso non ricordare i provvedimenti sull'occupazione per favorire le assunzioni a tempo indeterminato

In questi giorni, il nostro Governo sta lavorando in Europa per affermare definitivamente nei fatti che la crescita e l'occupazione sono la nostra priorità assoluta e che la flessibilità di bilancio può rappresentare un valido strumento per conseguire maggiore crescita e stabilità finanziaria. intende predisporre una manovra finanziaria coraggiosa e determinata, che coniughi l'esigenza della crescita con quella della tenuta dei conti pubblici (il sentiero stretto di cui si è parlato). Il cuore dell'agenda del Governo si concentra su un forte sostegno all'occupazione giovanile e ai motori della crescita, con la riattivazione degli investimenti pubblici, oltre alla riduzione delle disuguaglianze, nonché agli investimenti privati. Questo è il punto: i nostri sforzi oggi devono andare verso tutto ciò che può far crescere l'economia, creare il lavoro e rafforzare la coesione sociale. Partiamo da una buona base, ma è tempo di concretizzare nella legge di bilancio gli ultimi interventi di questa legislatura per dare alla crescita occupazionale ed economica una prospettiva più forte. Solo così l'Italia può ritrovare la strada giusta, indispensabile per rimanere fra i Paesi guida e per garantire un futuro migliore alle nostre imprese, ai nostri cittadini e alle giovani generazioni. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico ai provvedimenti di rendiconto e di assestamento.

Il problema è anche, e soprattutto, che con siffatta decisione è stata ancora una volta calpestata la dignità di questa istituzione. È stata calpestata la dignità della politica e anche dei suoi rappresentanti. Signora Presidente, per i comuni cittadini, ottenere una pensione quando non vengono rispettate le regole è impossibile. Per la casta e per qualcuno dei suoi rappresentanti, invece, pare si possano tranquillamente piegare a proprio piacimento le norme per avere, evidentemente, un ingiusto vantaggio, anche ricorrendo ad artifizi e raggiri. Ricordo che la lettera inviata dal senatore Cuomo al Senato riporta in maniera chiara e incontrovertibile la sua volontà di optare per il ruolo di sindaco e, quindi, di decadere da quello di senatore. Letteralmente egli ha scritto: «Il sottoscritto cessa da funzione e carica di senatore».

Non dia anche lei il suo contributo a umiliare ulteriormente questa istituzione. Altrimenti, lasceremo agli atti che si può conferire un vantaggio ingiusto a un parlamentare, piegando la legge a suo esclusivo vantaggio, e non perché ne abbia diritto, ma perché ha in tasca una tessera - guarda caso - del partito di maggioranza nel nostro Paese.

i colleghi del Movimento 5 Stelle, invece di occuparsi dell'ordinanza del tribunale di Palermo sulle loro irregolarità e sui loro comportamenti, spostano spostano l'attenzione su una situazione assolutamente legittima e corrispondente agli interessi di questa Assemblea e del collega Cuomo, come di tutti noi.

hanno risposto che, in qualunque modo noi oggi avessimo votato, anche se avessimo acceduto alle proposte del Gruppo del Movimento 5 Stelle, la procedura sarebbe comunque continuata per un numero di giorni tale da superare la fatidica data del 15 settembre.

non scaldare gli animi, che già sono caldi.

e, quindi, di far votare il Senato perché subentrino altri colleghi, in modo che loro non ne possano beneficiare. È semplicissimo.

costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Pagliari, se intende integrare la relazione scritta.

Non la butto fuori, ma la prego di rispettare le regole. So che le piacerebbe e invece niente. Deve rispettare le regole stando in Aula. *(Applausi dai in data 13 dicembre 2016 il tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, per accertare se la condotta oggetto del procedimento integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 22 dicembre il 22 dicembre 2016 e l'ha annunciata in Aula il 10 gennaio 2017. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 gennaio, del 1° e 22 febbraio e del 28 marzo Il senatore Gasparri è stato audito nel corso della seduta del 1° febbraio 2017 e ha fatto pervenire una memoria in data 9 febbraio 2017. In data 25 maggio 2016, il senatore Gasparri pubblicava sulla rete Twitter, attraverso il suo *account* @gasparripdl, in risposta a una utente della medesima rete, un commento del seguente tenore letterale: «Esempio di scuola

In data 12 luglio 2016 il signor Casaleggio ha sporto denuncia-querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona nei confronti del senatore Maurizio Gasparri; il procedimento è stato quindi trasmesso per competenza territoriale alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Quest'ultima ha trasmesso gli atti - avvalendosi della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 al tribunale di Roma, sezione del giudice per le indagini preliminari, il quale ha rilevato che si tratta di dichiarazioni *extra moenia* da sottoporre alla Camera di appartenenza per le valutazioni in ordine alla riconducibilità delle stesse alla previsione di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione. In tema di insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia*, la Corte costituzionale ha ormai un orientamento consolidato, in virtù del quale l'insindacabilità va riconosciuta in presenza dei presupposti di seguito indicati, il primo dei quali inerisce al nesso funzionale con l'attività parlamentare. richiesta in particolare una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possono collocarsi. Il secondo presupposto riguarda la ragionevole contestualità, ossia la dichiarazione *extra moenia* non può né precedere quella *intra moenia* (cioè l'opinione espressa nelle forme tipiche parlamentari), né essere dalla prima molto distanziata sul piano temporale. Infine la Corte costituzionale richiede l'identità soggettiva, ossia tutte le dichiarazioni devono essere dello stesso parlamentare. In ordine alla ragionevole contestualità, le date dell'atto ispettivo e del successivo *tweet* del 25 maggio 2016 evidenziano la ricorrenza di questo presupposto nel caso in esame. Parimenti è a dirsi per l'identità soggettiva: entrambi gli atti, infatti, sono stati compiuti dal senatore Gasparri. Relativamente al nesso funzionale, è necessario verificare il ricorso di una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio della funzione e gli atti esterni. Il *tweet* che ha originato la querela di Casaleggio Davide, in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione La struttura logico-giuridica della frase incriminata lascia spazio a due possibili interpretazioni. Da un lato, infatti, si potrebbe ritenere che la frase medesima sia costituita da due parti, che, pur se correlate, abbiano due diversi destinatari: la Casaleggio Associati Srl quanto a «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:» e la signora Silvia G. quanto a «Siete sterco @Silvia G.». Questa tesi trova un perno di appoggio nei due punti, che creano un'oggettiva cesura tra le due parti della frase, pur se la seconda persona plurale può essere un'oggettiva controindicazione In quest'ottica, l'unica frase di presunta lesività per la Casaleggio Associati Srl sarebbe la prima: «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:», essendo in ogni caso esclusa la lesività "in proprio" per il querelante per il noto principio dell'autonoma soggettività delle società a responsabilità limitata, persone giuridiche, rispetto a quella dei legali rappresentanti, persone fisiche, ed essendo la frase chiaramente ed esclusivamente riferita alla Casaleggio Associati Srl. Dall'altro lato, l'uso della seconda persona plurale potrebbe far ritenere la frase unica e non scindibile, avente come destinatari tanto la Casaleggio Associati Srl quanto la signora Silvia G. La comprovata esistenza di quest'ultima, però, è un oggettivo ostacolo a questa seconda interpretazione, imponendo di partire dalla prima interpretazione. In questa prospettiva, di conseguenza, la presunta lesività per il querelante è costituita dalla prima parte parte del *tweet* («Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:»), direttamente ed esclusivamente riferita alla Casaleggio Associati Srl e ai metodi dalla stessa adottati. Ciò premesso, si rileva che il *tweet* contestato esprime una critica che riguarda la scelta di fondo («offendono le persone»), la strategia comunicativa conseguente («non accettano la verità») e la preordinazione dell'attività della Casaleggio Associati Srl alla battaglia politica, condotta con dispregio di regole etiche e giuridico-costituzionali. In sostanza, il senatore Gasparri contesta alla Casaleggio Associati Srl la strategia della macchina del fango, tesa a screditare le persone, con mancanza di ogni rispetto delle stesse e della verità, dalla quale si prescinde volontariamente. Ed è una critica chiaramente rivolta alla Casaleggio Associati Srl sul presupposto, poi rivelatosi errato, che Silvia G. fosse un falso *account* e che, quindi, la persona non esistesse e che si trattasse di un nome inventato. Il che è come dire che il *tweet* del senatore Gasparri è rivolto alla Casaleggio Associati Srl, ai suoi metodi, alla sua attività politica, al suo modo di interferire nei sistemi di comunicazione, nella corrispondenza tra parlamentari e cittadini, con rischi per la libertà delle opinioni. Se così è, la sostanziale corrispondenza di significato, postulata dalla Corte costituzionale,

intenzione di ribadire una precedente convinzione: per l'appunto quella esposta nell'atto ispettivo *de quo*, nel quale vengono messi sotto accusa il ruolo della Casaleggio Associati Srl, i suoi metodi e la tendenza ad interferire nell'interlocuzione sui *social* con le *chat* telefoniche attenzionate, o gli audio corsari Il quadro di sintesi delle affermazioni, contenute nell'atto di sindacato ispettivo del senatore Gasparri, delinea la Casaleggio Associati Srl come una vera e propria struttura tesa a controllare l'informazione del M5S, ad orientare, di conseguenza, la comunicazione in chiave strumentale, cioè a fini politici. Che tutto questo sia giusto o sbagliato non è questione di competenza della Giunta, ma sul piano logico-giuridico è evidente la continuità con il *tweet*, che concretizza la sostanziale corrispondenza di significato indicato dalla giurisprudenza Da un lato, infatti, il senatore Gasparri parla di «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:», e l'atto di sindacato ispettivo illustra metodi, indirizzi di attività e strumenti usati di attività e strumenti che sinteticamente possono essere indicati con l'espressione, in chiave polemica e sintetica, di «scuola @casaleggio». Sulla base di queste conclusioni, si rileva che, pur ritenendo l'espressione «siete sterco» certamente inaccettabile, non verrebbe meno, in ogni caso, al di là dell'espressione colorita utilizzata, la corrispondenza sostanziale di significato, perché non potrebbe non ritenersi tale espressione come un apprezzamento meramente confermativo dell'accusa principale e comunque a essa strettamente collegato, con il conseguente permanere del requisito della sostanziale corrispondenza di significato. Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

per le argomentazioni del relatore, che non solo hanno una piena affidabilità giuridica sul metro delle tre tipologie segnalate dalla Corte costituzionale, ma riescono anche a onorare l'elemento irrinunciabile di ogni parlamentarismo: la libertà di opinione. Da questo punto di vista, siamo grati al collega e ci riconosciamo nella proposta della Giunta. Presidente, ci aspettano ancora lunghi mesi di dura campagna elettorale e sarà magari quella l'occasione per approcciarsi a uno degli appuntamenti politici forse più importanti degli ultimi decenni in Italia. Abbiamo compreso bene che quello che ci aspetta è quanto stiamo vivendo in ambito mediatico, comunicativo e politico già da tempo nelle Aule parlamentari.

quindi nella libertà di poter sostenere qualsiasi tesi e sapendo di non doverne rispondere in alcuna sede, se non, teoricamente,

la sedicente Beatrice Di Maio era in realtà la coniuge dell'onorevole Brunetta e ciò rende tutta la faccenda abbastanza ridicola. Ci sarebbe da sorridere. Il senatore Gasparri ha presentato un'interrogazione parlamentare sostenendo che, all'epoca, fosse opportuno indagare

sulla diffamazione, che rimarranno libere di scrivere qualsiasi fesseria e falsa notizia, sapendo di non doverne rispondere a livello civile e penale e neanche in via di autoregolamentazione della stampa. Bene, il messaggio che passerà sarà il seguente: presento un'interrogazione, invento uno scenario assolutamente fantasioso, sapendo che poi la cosa sarà ben pompata dalla stampa; dopo di che, su una piattaforma *social* come Facebook o Twitter

che si rappresenterà tra poco sarà questa realtà. Gli strumenti sacrosanti che la politica e i sistemi democratici parlamentari hanno costruito,

dal Gruppo M5S),* quella che sta aumentando l'astensionismo, quella che rende sensibili le pance di parte del Paese ai messaggi semplificati e veramente demagogici. L'antipolitica siete voi il Movimento 5 Stelle voterà contro la proposta della Giunta.

criticare. Possiamo semplicemente deplorare l'uso di un certo linguaggio, ma, nella fattispecie, mi pare assolutamente che si tratti di un caso che rientra nell'ipotesi di insindacabilità, trattandosi di una frase inserita in un contesto ben diverso. È stato già spiegato che gli interlocutori erano due non si può fare una valutazione estrapolando una parola o una frase rispetto a tutto il contesto che ha visto un dialogo prolungato nel quale il senatore Gasparri è stato più volte fatto oggetto di numerosi insulti e di altrettante offese. offese. Di tutto questo si è tenuto conto nella valutazione. E pensare o solo ipotizzare che qualcuno di noi parlamentari presenti delle interrogazioni preordinandosi l'idea di insultare qualcuno mi sembra davvero fantascientifico ed è addirittura ingenuo affermarlo. Credo che abbiamo prima di tutto il dovere del rispetto delle regole, che tante volte sono state richiamate. Bene, proviamo ad abituarci tutti a rispettare le regole, a partire dalle norme imposte dalla Costituzione, alla quale tutti abbiamo prestato giuramento. Dovremmo abituarci, forse, a rispettare di più quel contenuto, salvo che poi non decidiamo di cambiarlo, ma per farlo dobbiamo seguire ancora una volta le regole e la procedura.

Signora Presidente, colleghi, non volevo intervenire su questo punto, ma quanto detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, e in particolare dal collega Buccarella,

Ora, l'articolo 68 della Costituzione copre totalmente le opinioni dei parlamentari sia in sede parlamentare che esterna, le affermazioni che questi fanno si riferiscono all'attività politica ed è evidente che il contenuto degli interventi del collega Gasparri era in riferimento a situazioni specifiche e a situazioni generali che lo legittimano alle espressioni che lui ha formulato. Può aver usato un tono forte,

credo che debba finire questa storia per cui i colleghi del Movimento 5 Stelle in Aula possono interrompere chiunque, mentre ogni volta che parlano loro, se qualcuno li interrompe, loro manifestano in maniera intollerante.

è stato scritto, corredato da tutti gli insulti che abbiamo ricevuto, non soltanto io, ma tutti quelli che vengono definiti dissidenti, espulsi, rimossi,

con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri

reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli per il reato di cui

costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Augello, se

in circostanze di questo genere, il principio di insindacabilità previsto dall'articolo 68 della Costituzione. Infatti, il 7 marzo 2017 ci sono giunti gli atti relativi ad una querela per diffamazione inoltrata ai colleghi Mirabelli ed Esposito da un cittadino, il dottor Schiavone. La questione è molto semplice: in un *tweet* e poi successivamente in una conferenza stampa, secondo il querelante i due colleghi si erano resi responsabili del reato di diffamazione, accusando alcune associazioni, e in particolare quella del cittadino querelante, di non essere delle vere associazioni antimafia ma anzi di fare, direttamente o indirettamente, consapevolmente o inconsapevolmente, il gioco della mafia, delegittimando chi la combatte. Questo era l'oggetto della querela.

In particolare, abbiamo la seduta di Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, la n. 122 del 19 novembre 2015, in cui vi è una dichiarazione del senatore Esposito che va esattamente nella direzione delle affermazioni citate nella querela e che va poi letta integrandola con una lettera, anche questa agli atti della Commissione antimafia, che parlava esattamente dei problemi relativi ad un certo tipo di attività di alcune associazioni che si autodefiniscono antimafia e che, secondo il collega, non lo sono affatto.

abbiamo tutti gli elementi richiesti dalle varie sentenze della Corte costituzionale sia dal punto di vista temporale, perché tutti questi eventi (il *tweet* e la conferenza stampa) essere senz'altro considerati come un momento divulgativo delle posizioni assunte in Parlamento, sia perché tali posizioni sono state evidentemente assunte precedentemente nella medesima sede. Per tutte queste ragioni

il nostro Gruppo voterà a favore delle conclusioni della Giunta, abilmente sintetizzate dalla relazione del collega Augello.

per giustificare poi un atteggiamento e una evidente opera di diffamazione nei confronti di un soggetto terzo. Ora, io non mi dilungherò molto nei dettagli. Chiedo semplicemente ai colleghi che facciano come regolarmente questo Gruppo parlamentare ha fatto. Infatti, a differenza di quanto il vostro ex Presidente del Consiglio, oggi segretario del vostro partito, continua ad affermare,

privilegio in ambito processuale e ha chiesto di essere processato; processo che ovviamente, come era prevedibile, è andato in archiviazione. questo è quello che ritengono anche i senatori Esposito e Mirabelli, come qualunque altro cittadino si sottopongano al giudizio e al confronto con l'altra parte davanti a un giudice terzo e non vi si sottraggano, fruendo di questa impunità che ormai è diventata un privilegio di cui abusate in continuazione.

dagli elettori alla fine del suo mandato e a non dovere temere di spendere più di quello che gli viene dato per pagare gli avvocati e affrontare le cause giudiziarie quando denuncia ciò che ritiene

avvenuto nei casi che stiamo esaminando oggi, senza dover misurare le sue parole e sentirsi in imbarazzo se decide di chiamare «ladro» qualcuno che ritiene ladro, se decide di chiamare «profittatore» chi ritiene sia profittatore o se decide di dire che un certo gruppo di interesse,

che può permettersi di fare una causa ogni volta che qualcuno lo disturba, questo non vale per un parlamentare. Ecco perché è necessaria questa tutela e se c'è una parte che è intollerante e che a ogni insulto denuncia e porta in tribunale gli altri, non può questa parte avere la meglio su un parlamentare

alcune parole gentili con le quali il signor Beppe Grillo, *leader* del Movimento 5 Stelle, ha definito avversari politici - a volte parenti di avversari politici - una nostra collega a vita centenaria e un altro importante

vuol dire che andassero bene. Se si scambia la tolleranza, l'accettazione di un agone politico nel quale se ci si entra può capitare di essere attaccati (succede a ciascuno di noi), a ciascuno di noi), per acquiescenza allora non si è entrati nello spirito con il quale è stata scritta tutta la nostra Costituzione e, in particolare, l'articolo 68, una parte del quale resta ancora in vigore a tutela dei parlamentari che hanno il coraggio di dire ciò che pensano. Di questo coraggio c'è bisogno in ogni caso perché mettersi contro certi interessi può essere pericoloso, al di là delle sanzioni giudiziarie. giudiziarie. Un parlamentare che dice che una certa persona, un certo gruppo o una certa entità va contro gli interessi del Paese deve aver solo paura del giudizio degli elettori, di qualche vendetta tutt'altro che giudiziaria - cosa successa nel passato: alcuni politici hanno pagato molto caro e direttamente per aver toccato degli interessi troppo grandi - ma non di trascorrere il tempo in tribunale e di dover pagare

scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli

Signor Presidente, seppure in sintesi, in quanto la relazione completa è depositata agli atti di quest'Aula e quindi consente a tutti i colleghi di prendere atto del contenuto più complessivo, alcuni elementi devono essere esposti. La senatrice Bonfrisco risulta indagata, unitamente a Gaetano Zoccatelli, in relazione ai reati di cui agli articoli 416, 318 e 321 del codice penale. Secondo il capo di imputazione provvisorio, la senatrice Bonfrisco, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, avrebbe indebitamente accettato la promessa, ricevendo per sé e per altri, denaro e altre utilità da Gaetano Zoccatelli,

fornendo appoggio politico allo stesso, al cui apice era il citato Zoccatelli. La richiesta di autorizzazione in esame concerne 21 conversazioni telefoniche registrate tra il 26 febbraio 2015 ed il 14 ottobre 2015 nell'ambito del procedimento penale n. 15396. Nel ricostruire la vicenda processuale, il giudice per le indagini preliminari premette che nell'ambito del procedimento originario, che vede il signor Gaetano Zoccatelli quale principale imputato, si procede per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di turbative d'asta, nonché per altri reati-scopo relativi alla turbativa, fra le altre, di due gare bandite dall'ente pubblico CEV per la fornitura di energia elettrica, oltre ad episodi di falso in atto pubblico afferenti ai verbali di gara. In estrema sintesi, espone il giudice per le indagini preliminari che Gaetano Zoccatelli avrebbe rivestito pieni poteri gestori sia nel consorzio, che indiceva le gare di appalto, sia contemporaneamente in un gruppo di imprese commerciali operanti nel mercato delle fonti energetiche, quali la Global Power SpA e la E-Global Service SpA. Viene precisato che il signor Zoccatelli nonché entrambe le società incolpate dell'illecito amministrativo dipendente da reato hanno definito il processo con applicazione della pena nel corso dell'udienza preliminare (sentenza passata in giudicato), mentre per gli altri imputati il processo di primo grado è in corso di svolgimento

protratte sino al 19 febbraio 2016. Sottolinea il giudice per le indagini preliminari che, nel corso di tali operazioni, «si sono registrate una serie di conversazioni, che si concentrano maggiormente nell'arco di tempo che va dal mese di giugno 2015 dalle quali si ricava come Zoccatelli Gaetano si prodighi per ottenere l'inserimento del CEV nell'elenco dei 35 soggetti aggregatori. Il giudice per le indagini preliminari sottolinea in particolare la rilevanza dell'annotazione del 20 ottobre 2015, con la quale la polizia giudiziaria, nel condensare il contenuto delle conversazioni intercettate, ha evidenziato che «le indagini focalizzate alla ricerca di elementi di conforto all'ipotesi investigativa a carico di Zoccatelli Gaetano e dei suoi più stretti collaboratori, via via che proseguivano, portavano a delineare il ruolo della Senatrice», la quale appariva non solo a conoscenza della commistione commistione di ruoli di quest'ultimo nel CEV, ma come «una stabile promotrice». A fronte dell'attività svolta si sarebbe riscontrato il conseguimento, da parte della senatrice Bonfrisco, di una serie di vantaggi, quali di un contributo a sostegno della campagna elettorale di un esponente politico nelle elezioni amministrative in Veneto e nel pagamento integrale di un soggiorno

la consapevolezza di quest'ultima delle anomalie costituite dalla commistione fra CEV ed imprese del gruppo di Zoccatelli. In relazione a queste ultime, in particolare, le conversazioni del 25 maggio 2015 e del 9 giugno 2015 apparirebbero rilevanti - secondo il giudice per le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari ritiene che le intercettazioni oggetto della richiesta abbiano carattere casuale in quanto le operazioni sono state autorizzate nei confronti di un soggetto diverso dalla senatrice Bonfrisco.

dell'emersione della circostanza del pagamento». Ai fini della valutazione della necessità dell'utilizzazione probatoria delle intercettazioni, viene rilevato che l'attività di interessamento che si assume aver costituito la prestazione dell'accordo corruttivo si sarebbe svolta per lo più con contatti telefonici da parte della senatrice e che dall'attività di intercettazione si sarebbero riscontrati anche i vantaggi conseguiti; si rimarca che i contatti sono avvenuti in periodo coevo all'approvazione di un emendamento corroborare investigativamente la circostanza della corrispettività fra attività della senatrice e vantaggi elargiti dallo Zoccatelli in modo diverso dall'utilizzo delle elencate intercettazioni Nel caso di specie non appare verosimile che il pubblico ministero abbia appreso del coinvolgimento nelle indagini della senatrice Bonfrisco ben sette mesi dopo la telefonata del 9 marzo 2015 (ossia con la comunicazione scritta della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015), essendo invece plausibile che la polizia abbia immediatamente informato per le vie brevi lo stesso in considerazione della rilevanza dell'intercettato,

per le indagini preliminari in ordine alle stesse va respinta. Relativamente alle intercettazioni in questione risulta inutile un esame alla luce del parametro della necessità dell'atto

di necessità deve considerarsi, per così dire, assorbito nella valutazione della non fortuità. Per i motivi fin qui esposti, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015, con riferimento al documento IV, n. 15. ulteriori considerazioni di carattere generale in materia di immunità parlamentari e di limiti alla giurisdizione penale. L'esposizione di questa valutazione è agli atti ma alcune questioni intenderei richiamarle in Aula perché deve essere chiara una presa di coscienza dell'Assemblea stessa rispetto a questi profili. A prescindere dai profili inerenti alle intercettazioni e alla richiesta di autorizzazione in questione, si ritiene utile soffermarsi, *ad abundantiam*, sulla circostanza che, nel caso di specie, il sindacato espletato dall'autorità giudiziaria sull'attività emendativa posta in essere in sede parlamentare dalla senatrice Bonfrisco costituisce un'indebita ingerenza in attività parlamentari poste in essere *intra moenia*, rispetto alle quali, peraltro, i voti e le opinioni espresse non possono formare oggetto di valutazione sotto il profilo penale. È significativo a tale proposito rammentare che, pur con riferimento ad ambiti tematici di diversa natura, la Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1996 ha rilevato

poste in essere in tali sedi, che implicano valutazioni di natura politica, insindacabili in quanto tali e necessariamente libere nei fini politici da perseguire. si evidenzia poi che la sentenza n. 390 del 2007 è chiara, nel senso che solo un rimedio interno al processo, o al limite un conflitto di attribuzioni, può sanzionare l'atto invasivo costituito dall'intercettazione captata nella consapevolezza della potenzialità di incappare nelle conversazioni La soluzione della presente richiesta non potrebbe, quindi, essere altra che la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Ma occorre invece porsi il problema se la Giunta e il Senato possono pronunciarsi con un diniego per difendere l'attività parlamentare tipica e da dove si desumano i confini dell'atto tipico. Il magistrato è vincolato dal tenore della legge n. 140 del 2003; l'articolo 3, letto sistematicamente, potrebbe prescrivere che il giudice sia tenuto - pur non condividendolo - a trasmettere alla Camera competente gli atti. Tale lettura contribuisce a far sì che la pregiudiziale parlamentare eviti a monte violazioni delle immunità parlamentari in sede giurisdizionale. Colleghi, l'esposizione sarebbe ancora lunga. Credo di aver posto la questione in modo tale da sollecitare il vostro interesse e in questo senso richiamo l'attenzione di quest'Assemblea non soltanto su questa vicenda, ma anche sulle altre vicende che hanno riguardato

Presidente, ho apprezzato, non poco ma molto, la relazione della Giunta perché è stata centrata la questione. La questione è appunto centrata sulla conversazione del 9 marzo 2015, che intercorreva non già

In questa telefonata, si fa riferimento all'assunzione di tale Roberta Ferrara, persona conosciuta e comunque vicina alla senatrice Bonfrisco. Questa telefonata, per la verità, non viene presa in considerazione dal pubblico ministero, perché quest'ultimo ritiene che non vi siano profili di rilevanza penale. Cioè la senatrice Bonfrisco riceve un favore da un direttore generale di una società,

testualmente che il tipo di rapporto intercorrente tra la parlamentare e il soggetto sottoposto a controllo non si manifestava, in occasione delle captazioni,

dalla senatrice Bonfrisco e che facevano riferimento a un favore che la senatrice Bonfrisco avrebbe ricevuto da questo signore, consistente nell'assunzione di persona vicina alla senatrice Bonfrisco, non hanno

ha detto bene la Giunta, ha scritto bene il relatore: una polizia giudiziaria che ascolta una telefonata di tal tenore, vogliamo immaginare che non l'abbia detto al pubblico ministero? Lo ha informato, eccome se lo ha informato. Voi forse, che non siete operatori della giustizia, non frequentate le aule delle procure e dei tribunali, ma i rapporti tra pubblico ministero e polizia che indaga sono di contatto quotidiano. Io non posso essere preso in giro da alcuno nel momento in cui mi si viene a dire che questa rilevante circostanza non era stata riferita al pubblico ministero. Il pubblico ministero non era soddisfatto di questa telefonata, che di per sé sola non poteva costituire un'ipotesi di delitto nei confronti della senatrice Bonfrisco; aveva bisogno di altro e quindi ha continuato con intercettazioni per mirare esclusivamente a poter contestare ipotesi delittuose alla senatrice Bonfrisco. Noi sappiamo quanto siamo "appetibili" "appetibili" per le procure della Repubblica: come sentono il nome di un deputato o di un senatore si eccitano e quindi con questa eccitazione vanno avanti ad indagare per le più varie ragioni. ammesso e non concesso che la senatrice Bonfrisco avesse collaborato per l'emanazione di un emendamento, su quest'attività

non ha rilevanza penale e quindi non ritiene di iscrivere la senatrice Bonfrisco nel registro degli indagati.

persone ancora presenti in quest'Aula). Noi in quei casi dobbiamo fare in modo che ci si fermi. Personalmente, il Gruppo con amarezza apprendendo un'attività di tal genere da parte della sua magistratura, della magistratura italiana, afferma con forza che non possiamo autorizzare l'utilizzo di captazioni telefoniche che non sono state correttamente e legittimamente raccolte dal pubblico ministero e per queste ragioni ribadiamo

Io non gli avrei dato nulla, anche perché di quella cosina che gli diamo veramente non sapranno cosa farsene, perché in quella telefonata intercettata del 26 febbraio non c'è nessun elemento di rilevanza penale. Pertanto, volete fare, fatelo, ma fin da ora in quest'Aula io grido dicendo che i fatti non penalmente rilevanti non possono essere oggetto di contestazioni per una persona che riveste un ruolo istituzionale nel Parlamento italiano.

non avendo null'altro da aggiungere se non che ribadire la mia assoluta sottomissione all'istituzione parlamentare e alla sua irrinunciabile autonomia. modo, intendo, voglio e devo portare il medesimo rispetto per l'autonomia dell'attività d'indagine della magistratura che si compie quando, nel rispetto e nei limiti dello Stato di diritto, chiunque può essere indagato.

la non occasionalità delle intercettazioni; sotto questo aspetto, anche formalmente, la concessione dell'autorizzazione alla prima intercettazione, che è l'unica che può essere effettivamente avvenuta per casualità,

l'attività emendativa, così come tutta l'attività parlamentare di ogni membro di questo consesso e della Camera dei deputati. Consentitemi, infine, una considerazione di carattere strettamente personale; inviterei tutti i colleghi a prendere il fascicolo e leggere le intercettazioni.

Quando ci sono però delle regole e il rispetto dello Stato di diritto si sopporta anche di non avere vantaggi per evitare che una sorta di cattiva abitudine possa indebolire gli istituti parlamentari, quel Parlamento di cui tutti quanti facciamo parte. *(Applausi dal mi verrebbe da iniziare il mio intervento con l'invito «venghino, signori, venghino, alla sagra dell'impunità». Oggi è la giornata dell'impunità. Dopo aver regalato l'opportunità al senatore Cuomo di poter fruire della sua pensione dopo quattro anni e sei mesi di mesi di lavoro incessante in quest'Aula - cosa che ovviamente provocherà l'orticaria ai molti cittadini che lavorano quarant'anni per poter avere uno straccio di pensione

di cosa stiamo discutendo adesso. Non stiamo discutendo della colpevolezza della senatrice Bonfrisco. sta discutendo di eventuali responsabilità della senatrice Bonfrisco. Stiamo discutendo dell'utilizzabilità o meno di intercettazioni che se effettivamente la senatrice Bonfrisco, come lei sostiene e ovviamente sosterrà nelle sedi giudiziarie, non ha alcuna responsabilità, non possono che portare un beneficio alla sua causa e non altro. Che cosa stiamo autorizzando oggi (perché già sappiamo cosa voterete)? Stiamo dicendo a qualunque delinquente

di ottobre, leggendo le trascrizioni delle ultime intercettazioni, emerge che forse - ripeto, forse, perché saranno i giudice a deciderlo - c'è un altro filone di indagine che riguarda i rapporti presunti tra la senatrice Bonfrisco e il signor Zoccatelli, che riguardano un'altra cosa. Viene quindi aperto un nuovo fascicolo di indagine. Alla luce delle nuove informazioni, le precedenti intercettazioni, che prima non avevano alcuna importanza ed erano abbandonate assumono un altro aspetto, in quanto forniscono elementi che, insieme alle ultime intercettazioni, fanno aprire un altro filone di indagine. Ripeto, non so come finirà a livello giudiziario, ma si tratta di un nuovo filone di indagine. Oggi i giudici ci chiedono semplicemente di poter utilizzare

come un giurista, ha detto che la prima telefonata è fuori da quel periodo e ha voluto concedere l'autorizzazione. Non potete continuare con la storia dell'impunità come se in questo Parlamento ci fosse una regola

Partiamo dal presupposto che qui stiamo parlando ancora una volta, per l'ennesima volta, come ho detto nel precedente intervento, dell'osservanza stretta del dettato costituzionale. Di questo stiamo parlando, di quello che prevede la Costituzione riguardo all'attività dei parlamentari.

la quale si è sottoposta immediatamente all'interrogatorio, confermando esattamente il contenuto preciso, «paro paro», come si dice, di tutte le intercettazioni telefoniche. Questo a significare che comunque la senatrice Bonfrisco non ha nulla da nascondere e che questo ramo del Parlamento non intende sottrarre alcunché al giudice che si sta occupando della vicenda, che ha già in mano in mano integralmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche in quanto oggetto delle dichiarazioni rese dalla senatrice Bonfrisco. Torno a dire che qui stiamo semplicemente applicando la Costituzione e abbiamo deciso di autorizzare

chi ascoltava era a conoscenza dell'identità di uno degli interlocutori, cioè della senatrice Bonfrisco, quindi abbiamo deciso di dichiararne l'inutilizzabilità. Questa è la vicenda.

oggetto di indagine avrà il suo telefono intercettato e le sue telefonate verranno tutte utilizzate; non possono essere utilizzati, in virtù del dettato costituzionale, i colloqui con un

che ostacoli l'attività d'indagine e l'attività conoscitiva rispetto a quei determinati fatti in questa vicenda. Qui non si copre nessuno, l'indagine va avanti ugualmente nei confronti degli eventuali responsabili, dei quali sarà la magistratura ad occuparsi. Qui parliamo d'altro ed è inutile continuare - insisto - per scopi meramente propagandistici ed elettorali, a mistificare la verità. Rispettiamo la Costituzione e proviamo tutti insieme a difenderla, perché questo è anche il nostro dovere ed è questo che dovremmo fare sempre non adattandoci alle esigenze del giorno.

per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015. *(Segue la votazione)*.

Signor Presidente, Carrara è una città decorata di medaglia d'oro al valor civile, terra che ha visto stroncare la vita di molte persone dalla furia nazi-fascista, quindi non è accettabile che in questo territorio qualcuno possa ostentare sfrontatamente la bandiera fascista della Repubblica Sociale Italiana, addirittura a due passi dal sacrario delle vittime dell'eccidio di Vinca, dove furono trucidate 173 persone inermi. Non si può accettare l'elogio ai carnefici che hanno insanguinato Carrara e l'intera Penisola. Per questo motivo oggi deposito un'interrogazione indirizzata al ministro Minniti e alla ministra Fedeli sul caso della bandiera fascista esposta dall'insegnante carrarese Manfredo Bianchi sul Monte Sagro e sul Monte Brugiana e invito tutti i colleghi che credono fortemente nei principi antifascisti a sottoscrivere la mia interrogazione e li ringrazio. Gesto intollerabile a cui si aggiungono le sue dichiarazioni in una trasmissione radiofonica a diffusione nazionale, in cui esprime ammirazione nei confronti di Mussolini, definito «il miglior statista italiano di tutti i tempi» e apprezzamento alla politica economica di Hitler. Tali atti risultano estremamente gravi perché a compierli è un professore di una scuola superiore che dovrebbe essere un modello per le giovani generazioni, ed è grave che anche un consigliere comunale di Carrara abbia avallato con la sua partecipazione questo gesto. Nella condanna dei crimini compiuti dai nazi-fascisti ci deve essere unità da parte di tutte le forze politiche. Il fascismo, come ricordava il deputato Giacomo Matteotti, non è un'opinione, ma un crimine. In attesa che la giustizia faccia la sua parte e che gli ispettori del Ministero dell'istruzione verifichino la situazione, suggerisco a chi ha innalzato la bandiera fascista sul Monte Sagro e sul Monte Brugiana di andare a leggere la storia dei venti mesi di occupazione nazi-fascista. Si accorgerebbe che i fascisti di Salò sono stati complici degli eccidi, delle devastazioni e dei saccheggi. Manfredo Bianchi descrive i militari di Salò come gli unici che avrebbero tenuto alto il nome dell'Italia dopo l'8 settembre. Niente di più falso. L'esercito nazista e l'esercito della Repubblica Sociale Italiana nel solo territorio carrarese si macchiarono di crimini efferati, attuando un'occupazione militare fatta di prevaricazioni, abusi e soprusi di ogni tipo contro la popolazione civile. Tra le terribili stragi che si commemorano ogni ogni anno nel Comune di Carrara si annoverano: gli eccidi di Castelpoggio (33 vittime), di Bergiola Foscalina (72 vittime) e di Avenza (11 vittime). È una tragica storia fatta anche di deportazioni di migliaia di giovani fatti prigionieri e costretti a raggiungere la Germania su vagoni piombati, giovani strappati dalle loro famiglie, madri rimaste senza figli, mogli senza mariti, figli che reclamavano i loro padri. Molti non fecero più ritorno a casa. Gli atti compiuti dal professor Manfredo Bianchi risultano dunque particolarmente gravi e lesivi della memoria e dei valori su cui si fonda il nostro Paese e la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e dal coraggio di quegli uomini che si opposero al nazifascismo. Invito pertanto i Ministri da me interpellati ad intervenire quanto prima su quanto ho denunciato nella mia interrogazione. In questo periodo storico è facile dimenticare le conseguenze di una deriva autoritaria ed estremista. Abbiamo il dovere nei confronti delle giovani generazioni di non abbassare mai la guardia ed evitare qualsiasi imbarbarimento culturale. Carrara, il Movimento 5 Stelle e l'Italia tutta non dimenticano. Attendo le firme dei colleghi. Signor Presidente, con il mio intervento vorrei richiamare l'attenzione del Governo in merito ad un episodio molto grave che è avvenuto la scorsa notte nel Comune di Saronno. Ben sei autoveicoli (praticamente il parco macchine del Comune di Saronno) sono stati dati alle fiamme nottetempo con un'azione che ha certamente carattere intimidatorio. Ho avuto modo di parlarne con il sindaco, che ha sporto ovviamente denuncia, e oltre allo sbigottimento dello stesso, dobbiamo registrare quello della città intera che resta attonita di fronte ad un episodio che non ha eguali in quella realtà. Ci troviamo di fronte ad un'azione contro l'amministrazione comunale di Saronno, e chi ovviamente la rappresenta, che deve essere oggetto della massima attenzione da parte degli investigatori e da parte del Governo affinché, nei tempi più brevi possibili, i responsabili di questo terribile atto di intimidazione siano assicurati alla legge e soprattutto perché (e questo lo aggiungo avendoci fatto una debita riflessione) tutte le circostanze che stanno attorno a questo episodio siano valutate per tempo. A Saronno già negli anni passati abbiamo avuto episodi di violenza e di forte intimidazione da parte dei centri sociali nei confronti del Comune e il dubbio che questi episodi possano essere ricollegati a questi fatti sorge spontaneo. Certamente, come dicevo, signor Presidente, noi chiediamo che il Governo si attivi in tutti i modi nella maniera più determinata, dando supporto con azioni investigative che impediscano che chi ha fatto questo gesto possa lanciare un messaggio di sfida alle istituzioni e possa avere la soddisfazione del terrore e della intimidazione nei confronti dei soggetti, in questo caso il Comune, che ne sono

l'amore non uccide. Qualche giorno fa la famiglia Durini denuncia la scomparsa di Noemi, una ragazza di sedici anni di Specchia, un comune di poco meno di 5.000 abitanti in provincia di Lecce. A nulla sono servite le febbrili ricerche nei giorni passati nei casolari abbandonati, nelle grotte, nelle strade sterrate, nei pozzi e nelle campagne del Paese. La giovane vita di Noemi, purtroppo, è stata interrotta. Oggi il suo corpo è stato ritrovato a Castrignano del Capo, in località San Giuseppe, in provincia di Lecce. Si tratta, a quanto pare, dell'ennesima e drammatica storia di violenza sulle donne perché i giornali ci dicono che Noemi non è caduta, non si è procurata da sola la morte, ma è stata uccisa da un ragazzo di diciassette anni, il suo ragazzo, che sembra abbia confessato l'omicidio. L'amore non uccide. Secondo le ultime notizie, infatti, gli investigatori sono stati portati sul posto proprio dal fidanzato, ora indagato, insieme al padre, per omicidio volontario. L'amore non uccide. Una vicenda di inaudita brutalità che lascia senza parole e che riapre una drammatica ferita. In Italia, ogni due giorni, una donna viene uccisa. Ogni anno si conta un elenco impressionante di aggressioni, persecuzioni, maltrattamenti e abusi di ogni tipo. Numeri che fanno impressione, soprattutto perché, nella maggior parte dei casi, il nemico si trova tra le mura domestiche, tra quelli che dovrebbero essere i propri affetti. L'amore non uccide. Noemi, piccola ragazza dai mille sogni, non tornerà più a scuola, non uscirà più con i suoi amici, non valicherà i traguardi e le difficoltà della vita, perché la cieca violenza ha prevalso su tutto, scavando un solco doloroso. L'amore non uccide. Alla famiglia di Noemi, ai suoi amici e a chi le voleva davvero ben va il nostro abbraccio e il profondo cordoglio. Oggi si è scritta un'altra tremenda pagina di odio e prepotenza. L'amore non uccide.

Riteniamo questa nomina non adeguata e molto discutibile, sia nella scelta che nel tempismo, poiché la dottoressa Di Francesco dovrebbe andare in pensione a maggio 2018 e questa nomina sembra un regalo di fine carriera per una dirigente che, a nostro avviso, non sembra essersi distinta particolarmente per le decisioni che ha preso nella sua carriera come direttrice regionale dei beni culturali. A titolo esemplificativo

Pare che la decisione dell'allora direttrice regionale Carla Di Francesco di non apporre un vincolo alla palazzina abbia permesso di radere al suolo questo bene architettonico di grande valore storico per fare posto a un centro commerciale che pare non sia mai stato realizzato. A Ravenna invece la dottoressa Di Francesco pare abbia preso unilateralmente la decisione di modificare il vincolo indiretto, già apposto dalla soprintendenza di Ravenna, che tutelava il bellissimo Palazzo San Giacomo di Russi, in provincia di Ravenna,

caso che stiamo seguendo dall'inizio di questa legislatura. Infine, la dottoressa Di Francesco avrebbe bypassato, con il medesimo approccio, il parere negativo della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano,

Quindi - e concludo, ma potrei enumerarne altri - la dottoressa Di Francesco sarebbe stata anche al centro di un'indagine attivata dalla Ragioneria dello Stato per 400.000 euro di fondi pubblici destinati al restauro del Duomo di Modena dopo il sisma che colpì l'Emilia-Romagna nel maggio del 2012, per aver spezzettato detti fondi pubblici e i relativi appalti.

siccome la situazione che ha portato le Ferrovie dello Stato e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a commissariare

titoli sui giornali nazionali. Credo che l'azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul tema delle sicurezza sulle linee regionali sia importante e che sia bene concentrarsi sempre su quanto accade, soprattutto nelle situazioni in cui sembra che i problemi non si riescano a risolvere nonostante l'intervento